link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

è stato fatto di tutto per mettermi a tacere ancora una volta, per impedire che potessi partecipare a questa discussione! *(Applausi dal *(M5S)*. Perché questo avete fatto con deliberata intenzione: impedirmi PD)*, perché voi, che avete visto le carte e conoscete bene la questione, avete ben presente

commessa in campagna elettorale da un candidato deputato del PD, che si è presentato ad un comizio affacciato ad un balcone con accanto un soggetto di peso nella storia criminale della Provincia di Enna: è questo che voi non volevate sentire. MANCONI che si chiama Giannitto, ha una fedina penale lunga una pagina e mezzo, come rilevano gli atti. Leggiamo Leggiamo negli atti del procedimento: pluripregiudicato, arrestato per porto abusivo di armi da fuoco e condannato; arrestato per traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti; arrestato insieme a uno dei trenta criminali mafiosi più pericolosi, il latitante Di Fazio, condannato all'ergastolo per omicidio di un servitore dello Stato. Questa è la gente che vi portate in giro nei comizi, sul palco del vostro comitato elettorale! Giannitto, proposto per la sorveglianza speciale, condannato per favoreggiamento del suddetto mafioso,

Abbiamo poi anche Giovanni Scaminaci, altro soggetto

c'è poi Massimiliano Scaminaci, considerato dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura a capo nella Provincia di Enna di un'associazione dedita a che cosa? Al traffico di droga e condannato a dieci anni, lui e altri due arrestati da poco: Antonio e Giuseppe Scaminaci. Siamo dunque a cinque membri della famiglia Scaminaci, che sono parenti della moglie di Giannetto, che fanno dentro e fuori dalle patrie galere e dalle aule dei tribunali per reati gravi. E che cosa fa la vostra candidata?

nelle aule dei tribunali perché in un Paese normale il vostro candidato sindaco dovrebbe rispondere delle sue frequentazioni.

direzione) che l'interrogazione sui fatti di Enna è stata presentata troppo tardi. Certo! Solo per trovare tutto questo materiale su tutte queste persone ci vuole un'indagine della DIA, non di un semplice parlamentare.

avete macchiato la nostra Costituzione con l'abuso che avete fatto degli istituti a tutela delle prerogative parlamentari. Ormai sono visti come un abuso e noi di questo abuso non ce ne vogliamo fare nulla. Io inviterò i miei colleghi a votare contro

vergognare! È inutile che ti sbracci, Cociancich, hai massacrato la Costituzione e per questo sarai ricordato, vergognati! Vai fuori

provo alcuna vergogna per le accuse che mi vengono mosse da gente che va in giro con queste persone e fa campagna elettorale abusando dell'immunità perché la vostra candidata, deputata e avvocato penalista sa bene che andare in giro con un pluripregiudicato non comporta alcun rischio perché non può essere intercettata. Ma noi siamo pazienti e sappiamo che la magistratura arriverà, arriverà anche ad Agira e arriverà anche qua, arriverà anche a

Signor Presidente, colleghi, come avete avuto modo di verificare, gli interventi del collega Giarrusso sono, dentro quest'Aula e fuori dall'Aula, un po' fuori tono, diciamo così. Detto questo, però, io credo che intanto si debba ristabilire un equilibrio tra le varie questioni.

dentro e fuori da quest'Aula, sono evidenti, sono chiare e sono quelle che sono comparse durante i comizi, sulla rete stenografici di quest'Aula come sono stati nei Resoconti di quest'Aula anche i fatti. Ricordo alla Presidenza - non a lei, presidente Gasparri, ma al presidente del Senato che ho inoltrato con altri colleghi una denuncia nei confronti di colleghi senatori che, all'interno di quest'Assemblea, hanno impedito l'esercizio di un diritto fondamentale per un Parlamento: quello di andare a votare;

costituzionali. Però - ripeto - c'è differenza tra parole e fatti. Le parole sono evidenti; i politici dovrebbero vivere dentro e fuori dall'Aula di parole e svolgere la loro funzione istituzionale, certamente evitando affermazioni offensive. Ma, colleghi, in quest'Aula ne abbiamo dovute subire di tutti i tipi, anche questa mattina.

colpire coloro che hanno fatto quelle affermazioni gratuite e indimostrate. Detto questo, signor Presidente, colleghi, credo che nell'ambito di chi svolge un'attività quale quella che noi dobbiamo

C'è un punto però, Presidente, che credo debba essere chiarito: se ho presentato un'interrogazione parlamentare su un argomento ho la copertura costituzionale, se non l'ho

firmato mozioni di tutti i tipi: mi potrei permettere di insultare chiunque, in base a questa interpretazione della Corte e in base all'interpretazione della Giunta sul caso al nostro esame. Credo invece, signor Presidente, che non possa essere così: o c'è libertà di insulto sempre o non c'è libertà di insulto mai. Non è che uno si può parare il posteriore

perché solo così c'è il libero esercizio della funzione politico-parlamentare. Se la critica non può essere dura, se la critica non può andare su di tono, il più delle volte rimane inosservata. Badate che c'è una giustificazione all'attività piuttosto piuttosto violenta dal punto di vista verbale dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ieri qui in quest'Aula si è fatto un dibattito molto serio sulla questione Berlusconi; ebbene, se leggete i giornali di oggi del dibattito vero non c'è una parola, tranne su un caso: le posizioni giuridiche che sono state espresse in quest'Aula ieri non sono comparse. I principi, cari colleghi, signor Presidente, vengono allora utilizzati a comodo dalla stampa, da quest'Assemblea e dalla Giunta: è una cosa inaccettabile. L'ho detto più volte in Giunta: non ci possono essere due metri e due misure. Il collega Giarrusso, come sempre, va su di tono, come ha fatto anche oggi, ma non per questo bisogna usare il metro della sindacabilità o dell'insindacabilità per punirlo di questo suo atteggiamento o per punire coloro che su queste questioni eccedono di tono. È invece diversa la questione quando mi viene impedito di esercitare il mio diritto di voto, cosa che - ribadisco - è stata fatta in quest'Aula e alla denuncia della magistratura, con la copertura del Presidente del Senato, non c'è stata alcuna risposta se non quella dell'acqua fresca dei provvedimenti disciplinari. Per queste ragioni, signor Presidente, io sono per dare l'insindacabilità al collega Giarrusso, sia che lui l'abbia chiesta sia che non l'abbia chiesta, ma lui l'ha chiesta, perché agli atti della Giunta c'è la sua memoria in cui dice: io sono innocente. E probabilmente il collega Giarrusso lo è anche.

Signor Presidente, il mio Gruppo in quest'Aula voterà secondo la coscienza di ciascuno.

è materia così delicata e attiene alle posizioni personali di ciascun senatore che non può avere un'indicazione di partito. Ieri mi sono avvilito, per la verità, quando ho visto che i Gruppi parlamentari, anche in voto segreto, hanno votato grosso modo compatti, ora nell'una, ora nell'altra direzione. Personalmente, anche questa mattina per quanto riguarda il senatore Giarrusso, mi sono permesso di parlare con il mio Capogruppo, senatore Barani, per dare un'indicazione di voto che sia libero e rispondente alle emozioni della propria coscienza. Senatore Giarrusso, io voterò per l'insindacabilità, perché vede, senatore, credo di poter condividere quell'orientamento, anche sostenuto dallo stesso Senato nelle sedi giurisdizionali, secondo cui il concetto di insindacabilità deve essere interpretato nella maniera più estensiva possibile. attiene, per quanto mi riguarda, non già ad una prerogativa, ma ad una libertà di espressione di una critica politica, che talvolta può anche sconfinare in dichiarazioni che possono avere anche i toni ora dell'offesa, ora comunque di fatti penalmente rilevanti; ma ciò che per me ha importanza è lo spirito con il quale si pronunciano determinate frasi e dichiarazioni, ancorché esse possano ledere la dignità e la personalità di altri. Il senatore Giarrusso ha usato espressioni - come diceva il collega Buemi - dai toni forti, ma il senatore Giarrusso usa sempre i toni forti; dovrebbe finire sotto processo, allora, ogni qual volta usa toni forti, ma non mi pare che che il tono forte sia una fattispecie di delitto per la quale si può essere giudicati ed eventualmente condannati. Peraltro, non sono d'accordo con quell'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale la Giunta del Senato deve attenersi semplicemente, in maniera molto limitata e ristretta, a verificare se vi è o o no un'attinenza con l'attività parlamentare delle condotte dei singoli senatori anche fuori dall'Assemblea. Non sarei molto d'accordo neanche su questa perché un minimo di esame sulla fondatezza dell'accusa, a mio avviso, deve essere fatto, e nella fattispecie mi pare di potere condividere

hanno riportato sentenze di condanna, tanto che costoro non lo hanno querelato: se costoro lo avessero querelato, probabilmente Giarrusso avrebbe potuto dimostrare che la sua affermazione era corretta, perché c'era effettivamente una sentenza di condanna;

ancorché non commette reati, comunque si espone alla critica politica ed è ciò che ha fatto Giarrusso: ha criticato politicamente la vicinanza di un vicinanza di un politico con soggetti che documentalmente risultano essere responsabili di reati gravi e in particolare di mafia. Concludo, quindi, signor Presidente,

intimità della persona e in futuro non vi lasciate suggestionare ancora da principi rigidi ai quali talvolta mostrate di essere vincolati. Io mi auguro che questa mia dichiarazione, questo mio suggerimento e questo mio voto possano essere una affermazione di principi di garanzia e di tutela del Senato, ancora una volta anche in questa giornata, ma possano essere anche - ed è ciò che per me ha la rilevanza e l'importanza maggiori - una lezione di stile e di comportamento anche per i colleghi del Movimento 5 Stelle.

innanzitutto vorrei chiarire all'Assemblea che se siamo qui, è perché il collega Giarrusso lo ha chiesto esplicitamente: siamo qui perché il collega Giarrusso, in un atto giudiziario, ha chiesto che il suo procedimento venisse interrotto e fosse l'Assemblea del Senato a stabilire la sindacabilità delle sue affermazioni.

Detto questo, però, richiamerei l'Assemblea a una coerenza di comportamento, secondo la quale, come ha votato ieri per l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Stefano

Al collega di AL-A dico che se quello che ha detto il collega Giarrusso fosse confermato, costerebbe a quella collega qualche anno di carcere, perché il senatore Giarrusso non ha fatto un'affermazione generica, ma ha detto (e poi ha scritto) che la presenza di un mafioso sul balcone era

verrebbe arrestata, incarcerata e condannata, come è successo ad altri nostri colleghi in quest'Assemblea. Mettetevi allora nei panni di una candidata sindaco o di una parlamentare cui venga attribuito il fatto di di coprirsi con dei mafiosi per prendere voti e quindi di violare il codice penale: è evidente che deve reagire, non può far finta di non sentire. Le viene detto: «Lei viene eletta con i voti della mafia, lei esibisce il mafioso per intimidire la gente» e non reagisce? È evidente che deve difendere la sua onorabilità e querelare.

anche il senatore Stefano Esposito, nel momento in cui, come assessore, offendeva gravemente la reputazione di tre cittadini dirigenti avrebbe dovuto risponderne nel processo.

quest'Assemblea. Quando gli storici e gli studiosi andranno a vedere in questa legislatura - tra l'altro presieduta da un illustre magistrato - il tipo di giurisprudenza che viene portata avanti dalla Giunta, scopriranno che la convenienza prevale sempre sulla giustizia e su principi generali. L'ho detto ieri e lo ribadisco. Io, come il senatore Buemi, ritengo che quando un parlamentare, in Aula o fuori dall'Aula

metri fuori dall'Aula, magari commentando un colpo di Stato, il fatto di Vienna o una strage come quella di Nizza, in quel caso l'opinione politica è sindacabile. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Occorre sempre difendere il diritto del parlamentare ad esercitare la sua funzione;

Non possiamo dire, ieri, che è insindacabile un'affermazione offensiva nei confronti di tre persone e dire, oggi, che è sindacabile perché riguarda un collega del Movimento 5 Stelle. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come è possibile che un organismo come l'Assemblea

perché la collega Greco ha il sacrosanto diritto di difendersi nel processo da accuse infamanti che le potrebbero costare il carcere o, comunque, una accusa gravissima nei suoi confronti come quella di voto di scambio mafioso.

Presidente, mi ha fatto molto piacere che le modalità del voto di ieri abbiano portato il senatore Giarrusso a esprimersi.

luogo, mi sembra che qui si tratti di lotta politica, una lotta politica i cui toni non condivido. Ma è lotta politica e, allora, mi sembra che l'insindacabilità sia sacrosanta. Dobbiamo ricordare,

In verità, il senatore Giarrusso aveva inizialmente chiesto l'insindacabilità in sede processuale, reiterando poi questa richiesta che avrebbe aperto, evidentemente,

poco prima di iniziare la discussione generale e di arrivare al voto il senatore Giarrusso ha manifestato, tramite un'agenzia di stampa (che peraltro è stata confermata dai suoi colleghi di Gruppo), la volontà di rinunciare all'insindacabilità, chiedendo che la Giunta si pronunciasse

a prendere posizioni ed esprimere scelte che non corrispondono al suo vero volere. Egli deve dire certe cose che non pensa in cuor suo. Se così non fosse, non saremmo arrivati a questo, come è stato segnalato anche dal collega Giovanardi.

una corrispondenza sostanziale di contenuto tra le opinioni espresse all'esterno e le opinioni espresse nelle Aule parlamentari.

permeato da un ipergarantismo che rischia di confondere i piani, perché il garantismo deve essere anche la garanzia delle libertà e dei diritti delle persone. Passiamo ai fatti. Il senatore Giarrusso ha reso affermazioni gravemente lesive

come tale e poter dimostrare che i fatti riferiti non sono veri. Se fossero veri, la magistratura avrebbe avuto gli elementi per archiviare e non procedere. La magistratura ha ritenuto

ha proceduto. Il senatore Giarrusso ha tentato di utilizzare in quel procedimento lo scudo dell'articolo 68 della Costituzione, quello scudo che il Movimento 5 Stelle ha sempre tacciato come privilegio della casta. Ha tentato reiteratamente di utilizzare quello scudo, e ha tentato di farlo con le sue memorie alla Giunta. Non ha mai rinunciato allo scudo, a cui non si rinuncia con un'agenzia Ansa,

questione relativa all'esercizio della propria funzione. Anche con un atto ispettivo si possono ledere la dignità e l'onore di una persona, la quale ha diritto a difendersi. La Corte costituzionale non dice questo. Dice che, per per valutare se ci sia l'attinenza, ci deve essere quantomeno l'atto di esercizio della funzione di parlamentare. In detto caso non c'è neanche questo. C'è stato il tentativo artificioso di coprire un fatto privato, un'accusa lesiva gravissima della dignità e dell'onore di una persona con un atto ispettivo depositato nove mesi dopo. *(Applausi dal

In premessa osservo che la richiesta fatta ieri dal senatore Giarrusso di essere presente durante la discussione che avrebbe portato al voto su una sua possibile insindacabilità non è stata parimenti avanzata in Giunta.

Se siamo per la difesa dei principi democratici e poiché tutti noi, da questa e dall'altra parte dell'emiciclo, sappiamo che il diritto all'insindacabilità è irrinunciabile, tant'è che lo votiamo,

dell'insindacabilità, delle disposizioni costituzionali e, quindi, dei principi democratici. Ma, ancora, due pesi e due misure sono usati perché il senatore Giarrusso, in Giunta, fa pervenire, per quanto discutibile rispetto ai principi democratici e costituzionali dell'irrinunciabilità, una richiesta di insindacabilità, mentre qui vi rinunzia - vi rinunzia - probabilmente anche a seguito di un *post* grillino messo su Facebook o in chissà quale sito - prima ancora che ci fosse la riunione, soltanto tre ore prima. Per cui in Giunta abbiamo avuto la sovrapposizione di una richiesta e di un annunzio via *web*.

deputata alla Camera, e un senatore della Repubblica che si sono scambiati, durante un'occasione elettorale, epiteti violenti e accuse reciproche.

oltre modo e ancor più rispetto a quello che sono, occupate nel dirimere contenziosi tra parlamentari. Mi sembra pruriginoso il fatto che il PD,

stamattina - abbia due pesi e due misure quando si parla di un suo parlamentare - come ieri è successo per il senatore Esposito, a seguito della mia relazione, che ha ricevuto 190 voti per l'insindacabilità come dichiara di volersi comportare nel caso del senatore Giarrusso. Il senatore Giarrusso, fra le altre cose, è difeso da una specifica deliberazione della Giunta, allorché si dice che, quando

attingere a toni assai marcati e coloriti. Ricordo che non stavamo in una piazza della Provincia di Bolzano! Stavamo nella piazza di una Provincia siciliana e quell'epiteto il senatore Giarrusso credo credo possa averlo contemperato nel normale dibattito politico che si ha a quella latitudine. Quindi, in ossequio ai principi ai quali si sono la Camera dei deputati e il Senato e alla giurisprudenza parlamentare, come ho fatto in Giunta, continuerò a votare per l'insindacabilità del senatore Giarrusso. E ritengo a questo punto, vista la sensibilità di tutti i componenti di questo augusto consesso, che dovremmo procedere per voto segreto.

non può dimettersi.

che propone di punire i sorvegliati speciali e i condannati per associazione mafiosa in modo da evitare che le istituzioni siano passibili di infiltrazioni malavitose. Io mi chiedo perché non sia stata sollecitata la sua calendarizzazione e non si sia provveduto, per coerenza. Detto ciò, faccio anche una battuta e chiedo: ma il senatore Giarrusso, di fronte a un tema così importante e così caro al Movimento 5 Stelle, quando quando ha risposto dando ragione all'indicazione del giudice, ha consultato la rete e il *blog*? Ha consultato i cittadini su cosa doveva o non doveva fare oppure ha agito di propria iniziativa, visto che dopo c'è stata una rettifica da parte di Crimi? Giarrusso potrebbe valere il discorso dell'insindacabilità, ma potrebbe essere soggetto passibile di espulsione dal Movimento 5 Stelle, coerenza per coerenza.

Non c'erano le prove, eppure potevamo dirlo, e ne avremmo giustamente dovuto rispondere nelle aule di tribunale. In sostanza, voglio dire che quando, nell'ambito delle nostre prerogative parlamentari,

potrà dare ragione allo stesso Giarrusso. Ma - ripeto - in quel caso che ho citato penso di non aver mai sentito alcun parlamentare esprimersi in certi modi nei confronti del direttorio, perché sono convinto che non era e non è vicino ad ambienti camorristici.

Se valutiamo queste dichiarazioni, possiamo allora affermare che il direttorio era vicino ad ambienti camorristici? Non penso. Quindi, il senatore Giarrusso, che - è vero - usa sempre toni accesi (e lo fa anche quando starnuta), ne risponderà in tribunale, dove si difenderà con un legale che lo assisterà e pagherà le conseguenze se quanto ha affermato

hanno posto la questione di dare all'insindacabilità una interpretazione estesa che vada al di là dei paletti fissati dalla Corte costituzionale. Lo stesso presidente Gasparri ha ricordato

che, dal punto di vista della Corte costituzionale, le norme, così come sono in questo momento, consentono il ricorso all'insindacabilità soltanto quando le esternazioni, le dichiarazioni *extra moenia*, siano un'amplificazione coerente e puntuale dell'attività parlamentare svolta *intra moenia*. Questo è un fatto. Quindi, nel momento in cui il relatore, chiunque sia, deve affrontare una materia di tal genere, non può prescindere da siffatta cornice.

esiste la possibilità che un parlamentare svolga un intervento *extra moenia* seguito a brevissima distanza da una dichiarazione in Parlamento. In quel caso si può a buon diritto ancora invocare l'insindacabilità. La fattispecie di fronte alla quale ci troviamo - come ho già detto nella relazione - è completamente diversa e quindi, doverosamente, chiunque si trovi a svolgere la funzione di relatore in casi come questi non può che tenere conto delle regole

Il senatore Giarrusso, oggi, ci dice - in maniera un po' tonitruante - che non ha alcuna intenzione di sottrarsi al giudizio di merito e, nella sostanza,

che in sede di replica diventa inevitabile, però, porre al senatore Giarrusso alcune domande molto semplici dal punto di vista proprio del relatore. Non

la domanda di fondo è la seguente: per quale motivo il 23 giugno 2016 e il 29 giugno 2016 è stato imposto un lavoro alla Giunta e al sottoscritto per verificare se i motivi dell'insindacabilità invocata da Giarrusso fossero fondati o no dal punto di vista giuridico e formale? Questa è una domanda importante, perché perché l'utilizzo del Senato della Repubblica come cassa di risonanza per mettere in evidenza la situazione di un territorio attraverso lo strumento del trascinamento in Giunta di un caso che, tra l'altro, risale al 2015 - quindi, aggiungiamo che la querela è ferma da più di un anno - è già ai limiti, ma non spetta a me giudicarlo.

quando e se avesse presentato la sua interrogazione e se fosse o no un motivo di insindacabilità; quando e se fosse effettivamente presente una scriminante dei suoi diritti diritti di esprimere le sue opinioni politiche; quando e se vi fosse un'insussistenza o un'indeterminatezza del destinatario delle sue accuse che oggi con chiarezza ci ha spiegato in Aula che pare non ci sia. sia. Questo elemento in sede di replica non posso non metterlo in evidenza, perché altrimenti, signor Presidente, sembriamo tutti matti. Sembrerebbe quasi che io abbia svolto una relazione perché mi sono inventato, o l'Assemblea si è inventata, una richiesta di insindacabilità, che invece è stata motivata, seppure

accusando il collega Giarrusso, che fosse un scudo per evitare il problema della querela. È il senatore Giarrusso che l'ha utilizzata come uno scudo spiegandoci che l'aveva presentata otto mesi dopo, altrimenti non l'avrei mai citata; mai mi sarei permesso e mai mi sarebbe venuto in mente. tutto questo non sia permesso. Per carità, Presidente, tutti ci possono ripensare e non c'è nulla di strano. D'altronde, da questo punto di vista non c'è giurisprudenza. C'è solo il Nuovo Testamento che ha perdonato San Pietro perché, per tre volte, ha rinnegato Gesù. Insomma, nel caso di specie, c'è almeno il numero tre come limite della possibilità di rinnegare qualcosa o di ripensarci. Il problema di fondo, però, è che credo, anche per la qualità del lavoro che dobbiamo svolgere in Giunta,

all'insindacabilità nel giorno stesso in cui se ne sta discutendo. È una questione formale, ma la forma è sostanza quando si tratta di un organismo delicato come quello che noi siamo chiamati a gestire per conto del Senato della Repubblica. Ed è una questione che inevitabilmente, in sede di replica, avevo il dovere di mettere in evidenza.

si atterrà alla libertà di coscienza. Per quello che mi riguarda, non intendo derogare al principio volteriano:

Se questo principio vale per tutti noi, deve valere anche per il senatore Giarrusso. Non c'è niente che colleghi una mia idea alle idee di Giarrusso. Sono stato forse tra i pochi qua dentro, nel dormiveglia generale, a contrastare un'opera di delegittimazione costante del Parlamento e dei parlamentari, a ribellarmi alle reiterate accuse, alle menzogne di volerci dipingere come una casta bieca e senza cuore, che vive di agi e di prebende, nel mentre il popolo viene affamato. Giarrusso è espressione di questo, è il segno dei tempi e, quindi, agisce nei confronti degli altri con il sussiego di una superiorità morale che non trova alcun riscontro. Agisce in maniera volgare, tracotante, e avrà fatto questo anche durante quel comizio. Egli elargisce patenti di democrazia, di onestà: «onestà, onestà, ta-ra-ta-tà» - conosciamo questa canzoncina - ma ha diritto di farlo, perché dovremmo contrastarli qua dentro i Giarrusso, ogni qualvolta mistificano la realtà, ogni qualvolta si ergono a depositari di una morale.

Ma difendo qua dentro il suo diritto a dire quel che deve dire, perché il mio voto contro la sindacabilità per Giarrusso non è una cortesia, ma il rinfaccio di un liberale a un farlocco giacobino.

Ho sentito il senatore Buemi parlare di insulti, ma qui non stiamo parlando di insulti. Ho sentito il senatore Carraro parlare di lotta politica, ma qui nessuno parla di lotta politica quando voi sostenete determinate cose. Ho sentito - e

parole. Il nostro collega è stato accusato da una vostra deputata e candidata sindaco del Partito Democratico, Greco Maria Gaetana, per aver detto: «È inammissibile, è intollerabile che nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in campagna elettorale». La vostra candidata sindaco nel Partito Democratico nonché deputata ammette la presenza su quel balcone di tale Giannitto, il quale, come abbiamo detto, ha una fedina penale abbastanza importante. Quello che voi dovreste dire e quello che noi chiediamo è semplicemente un fatto molto importante.

se poi domani sera un politico va a cena con quello che è andato a cena con Buzzi e Carminati, la mia morale mi permette di dire, tra virgolette, che anche io sono andato a cena con Buzzi e Carminati. Il sillogismo politico mi permette di dire che se c'è un Ministro che fa approvare emendamenti per il suo compagno e quel Ministro è del mio partito, allora anche io ho permesso di far approvare quell'emendamento. Questo è il sillogismo politico. Noi tutti sappiamo che quel tale Giannitto, pluripregiudicato, che stava sullo stesso balcone con un candidato sindaco del PD,

perché non è importante cosa è legale. Noi non siamo tenuti ad aggrapparci a quello che è legale,

voi pensate che il fatto che siete dotati di immunità parlamentare e di insindacabilità vi pone su un piedistallo di differenza rispetto agli altri cittadini; noi diciamo semplicemente…

ma stiamo per deliberare sulla sindacabilità o insindacabilità delle sue dichiarazioni, delle parole che ha pronunciato nel corso di un comizio. Una volta che il Senato viene investito di questo compito è su questo che deve deliberare. Poteva accadere che noi fossimo investiti di questo compito perché il giudice, direttamente, di sua iniziativa, senza che lo chiedesse nessuno, interpellasse il Senato per sapere se il Senato riteneva che quelle parole e quelle dichiarazioni facessero parte del compito di parlamentare, fossero quindi inerenti all'attività di parlamentare oppure no.

la richiesta del senatore Giarrusso era di archiviazione, ritenendo evidentemente che le sue dichiarazioni non fossero offensive e non costituissero comunque reato; in subordine, chiedeva di avvalersi dell'articolo 68 della Costituzione, ritenendo dunque le sue parole insindacabili in quanto facenti parte della sua attività parlamentare. Richiesta analoga è stata fatta nelle memorie scritte che il senatore Giarrusso ha presentato presso la Giunta delle elezioni

di cambiare il suo orientamento e il suo sentire rispetto a questa vicenda giudiziaria; potrebbe cambiare idea anche domani, dopo che quest'Assemblea si sia espressa. Ma noi non stiamo a giudicare sulla volontà del senatore Giarrusso di andare in tribunale a difendersi e ad agire in quella causa; stiamo giudicando se quelle dichiarazioni facciano parte di una attività politica oppure no. L'intervento del senatore Lucidi ha dimostrato chiaramente che si tratta di lotta politica, l'ha detto nel modo più chiaro possibile. l'ha detto nel modo più chiaro possibile. Si tratta, come ha detto il senatore Carraro, di lotta politica, fatta in un certo modo; lotta politica che il senatore Lucidi ha proseguito in questo intervento in Assemblea, attaccando tutti gli avversari e ascrivendo al proprio partito le somme virtù civiche. È un intervento politico, come politico era l'intervento del senatore Giarrusso. Poco importa che ora dicano «rinunciamo», «votate così» o «votate in quest'altro modo». Oggi

Pertanto noi, non giudicando mai su queste materie secondo l'appartenenza politica, dobbiamo chiederci se, in generale, una persona che ravvisi, a suo parere, contiguità da parte di certe persone rispetto ad ambienti criminali, vi sia il ambienti criminali, vi sia il diritto, da parte di chi viene colpito, di ribadire le proprie ragioni. Nel momento in cui il Senato viene investito di tale questione, deve giudicare se sia lecito fare politica in questo modo, senza fare nomi, accusando

serve a garantire che un parlamentare possa fare una lotta politica senza temere da parte avversa delle azioni giudiziarie estremamente onerose. E magari per la parte avversa queste azioni onerose non sono, perché la parte avversa è molto potente. Non mi riferisco, naturalmente a questo caso, ma noi dobbiamo riferirci ai casi generali. Per quanto noi voteremo contro la deliberazione della Giunta, ritenendo che oggi, come in tutte le altri occasioni (e non dobbiamo andare tanto indietro nel tempo), nel momento in cui un parlamentare conduce una lotta politica e rilascia dichiarazioni, e rilascia dichiarazioni, anche di pesante attacco politico, abbia il diritto di farlo senza temere conseguenze ingiuste

ha pronunciato quelle frasi? Perché stava tenendo un comizio politico. Non avesse avuto un ruolo politico, neanche sarebbe stato chiamato su quel palco. In questo modo noi non tuteliamo il senatore Giarrusso, il senatore Giarrusso, ma il diritto dei cittadini a essere rappresentati da persone che sono libere di svolgere un'attività politica, facendo anche delle accuse gravi, purché restino circoscritte all'aspetto politico.

perché si è sentita evidentemente toccata, ma consci che un parlamentare deve poter svolgere la sua attività in ambito politico senza che le sue accuse di carattere politico possano costituire un danno al suo patrimonio, alla sua onorabilità e alla sua fedina penale, noi voteremo

Signor Presidente, quest'Assemblea ci ha abituato, purtroppo, a interventi volgari, violenti, offensivi, ma non mi sentirei tranquilla con me stessa, come donna e come parlamentare, se non rilevassi il maschilismo e il sessismo becero dell'intervento del senatore D'Anna.

Mario Giarrusso ha ritrattato in poche ore la sua posizione. Sono stata in questo Gruppo e ho visto e so che cosa è la coercizione di un Gruppo

Voterei sì se fossi convinta che tu abbia assunto questa scelta in maniera libera, ma sono certa che tu questo non l'hai fatto. Per questo motivo, dichiaro il mio voto contrario.

nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Quindi, chi vota a favore riconosce la validità della proposta della non sussistenza dei requisiti, mentre chi vota contro ritiene che i

il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015». Noi tutti

in merito alla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, altresì definita e denominata legge di delegazione europea 2015, credo sia opportuno fare alcune riflessioni preliminari

Questo sta a significare che la relazione non è una semplice elencazione, ma una descrizione di tutti i vari aspetti che caratterizzano questa legge di delegazione europea

è stata caratterizzata non solo da approfondimento, ma da una pacatezza dialogica e da una dialettica che ha significato l'assunzione di grande responsabilità da parte della Commissione stessa, saggiamente presieduta dal senatore Chiti.

la nostra 14a Commissione), come un momento ulteriore di costruzione di quell'unità europea e di quella condivisione di valori dei quali, signor Presidente e signori colleghi senatori, oggi c'è assoluta necessità. La nostra azione, anche trattando questa tematica, non deve essere un'azione cosiddetta centrifuga, che caratterizza il dibattito a livello europeo, ma deve essere un dibattito centripeto,

un'ulteriore riflessione alla vostra attenzione, a mo' di premessa, perché sta a significare anche le modalità che caratterizzeranno i lavori delle prossime ore e dei prossimi giorni in tema di legge di delegazione europea. Sappiamo che il disegno di legge annuale di delegazione europea è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2016. Un successivo disegno di legge di delegazione europea quindi sarà presentato per l'anno 2016 e il Governo, nel corso dell'esame in 14a Commissione, si è impegnato a presentarlo in tempi rapidi, partendo nel suo *iter* legislativo proprio dal Senato stesso. È un disegno di legge abbastanza corposo, quello in esame, come modificato e approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di ben ventuno articoli e di due allegati. Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di tredici direttive, una decisione quadro, di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e di due direttive da attuare in via regolamentare, nonché delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a dodici regolamenti.

- che nel corso dell'esame in Commissione non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge. Ciò ha

Ciò in ottemperanza a specifiche intese intercorse con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e con il Governo, secondo le quali il disegno di legge di delegazione europea 2015, già approvato dalla Camera, avrebbe dovuto essere approvato dal Senato senza modifiche, mentre, reciprocamente, il disegno di legge europea 2015-2016, approvato dal Senato, non avrebbe dovuto essere modificato dalla Camera, come poi in effetti è avvenuto, con l'approvazione definitiva intervenuta il 30 giugno del corrente anno. Nel corso dell'esame in Commissione è stato peraltro concordato che eventuali questioni problematiche avrebbero potuto essere affrontate mediante la proposizione di puntuali ordini del giorno, di cui darò conto nel prosieguo della relazione. Va comunque sottolineato che, sin dall'inizio della legislatura, c'è stato un importante lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo nel recepimento delle direttive europee e nella sanatoria delle infrazioni. A tale lavoro ha fornito un indubbio supporto la legge n. 234 del 2012, che ha permesso di avere a disposizione non più soltanto l'unico strumento annuale della legge comunitaria, ma i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, suscettibili di essere adottate nuovamente nel corso dell'anno di riferimento, per un potenziale di ben quattro leggi di sistema all'anno per recepire il diritto dell'Unione europea. Inoltre, l'aver ripartito l'esame del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea tra le Commissioni affari europei di Senato e Camera, che quindi lavorano contestualmente e senza tempi di sospensione, con il vincolo politico che la Camera che esamina per seconda non apporta modifiche al testo approvato dalla Camera che esamina per prima, ha reso estremamente celere l'*iter* legislativo. evidente che la celerità dell'*iter* legislativo si è sostanziata e fondata anche sull'accordo e sul consenso di tutti i componenti dei vari Gruppi all'interno della 14a Commissione.

andando per sintesi su quegli articoli che non hanno subìto modificazioni alla Camera né hanno dato luogo alla presentazione e all'approvazione di ordini del giorno in sede di 14a Commissione del Senato. Quindi, sull'abbrivo di quanto accennavo poc'anzi sulla modalità espositiva da parte mia su questa relazione, sull'articolo 1 vado rapidamente a richiamare che reca delega al Governo per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B. L'articolo 2 reca delega legislativa in merito alle sanzioni penali o amministrative, per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa. Un approfondimento particolare merita l'articolo 3, che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in merito alla prevenzione, alla gestione, all'introduzione e alla diffusione di cosiddette specie esotiche invasive, nell'ambito del quale, nel corso dell'esame in Commissione, è stata approvato, come anticipavo, un ordine del giorno, in particolare l'ordine del giorno G3.100, con cui si impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene, provenienti dal traffico navale extra Mediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat*, delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'ecosistema marino. L'articolo 4 è stato introdotto dalla Camera durante l'esame del disegno di legge e porta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La Commissione europea a tal proposito ha archiviato, il 28 aprile 2016, la procedura d'infrazione 2011/4030.

sul quale si è dibattuto molto in Commissione, ma anche in Assemblea, alla luce di altri disegni di legge; un tema che vede l'Italia particolarmente interessata e coinvolta per ovvi motivi. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati due ordini del giorno. Il primo impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento del 2011 dell'Unione europea, al fine di garantire la corretta - questo è l'aspetto particolarmente significativo e importante importante - e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera agroalimentare in quanto importante a dare la massima trasparenza. E credo che questo risponda anche a criteri di eticità

che evidentemente l'attenzione è molto puntuale e precisa e che la finalità, appunto, è tutelare la salute del consumatore in merito all'uso di prodotti su cui il dibattito di queste ultime settimane,

del giorno G8.100 con cui si impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo da un lato che si realizzi un maggiore coinvolgimento delle imprese stesse nel processo di definizione della normazione e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico. L'articolo 9 richiama le condizioni da armonizzare per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'articolo 10 è relativo al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali ed in particolare dispone la creazione di un apposito comitato nazionale per le politiche macroprudenziali cui partecipano le autorità del settore bancario e finanziario. Il comitato, presieduto dalla Banca d'Italia, avrà specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazioni nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici nonché enti privati.

con il primo si impegno il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori. Con il secondo si impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità connesse all'attuazione della direttiva n. 59 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. del giorno impegna il Governo a prevedere che il comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo alcuni principi e criteri direttivi puntualmente indicati. L'articolo 11 si riferisce alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. L'articolo 12 è stato introdotto durante l'esame del disegno di legge servizi di pagamento nel mercato interno. Anche in questo caso la 14a Commissione è intervenuta con alcuni ordini del giorno e nel corso di questo esame ne è stato approvato in particolare uno con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale prevedendo, in particolare, questo è un dato che tengo particolarmente a sottolineare, una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi. È intuibile quali benefici se ne possano trarre, non solamente per quanto riguarda l'aspetto squisitamente bancario e finanziario, ma anche per quanto riguarda tutte le tematiche, facilmente immaginabili, ad esse connesse.

delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Anche in questo caso sono stati presentati due ordini del giorno: il primo (G14.100) impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92 dell'Unione europea sia previsto un sistema di tutela più ampio

affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

nell'ambito della suddetta direttiva, sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

15 è relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tema quindi di particolare importanza

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, tema ecologico di grandissima importanza e rilievo per tutte le ripercussioni che si hanno, non soltanto sotto il profilo produttivo ed energetico, ma ancor più sotto il profilo della L'articolo 17 si riferisce alla limitazioni delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Credo che questi siano temi di grandissimo rilievo e spessore a livello europeo

l'articolo 20, che è stato introdotto durante l'esame alla Camera e che si riferisce alla gestione collettiva dei diritti d'autore. Questo

possiamo definire *bipartisan* e trasversali che stanno a significare anche la modalità con la quale si è lavorato in Commissione. Infatti, un primo ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva; a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione - passaggio particolarmente significativo - ad altri organismi di gestione collettiva; collettiva; a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere

degli altri Stati membri dell'Unione europea e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal gruppo di esperti istituito dall'articolo 41 della direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

direi ancor più conflittuale e notevolmente critico, dove si sono messi e si mettono in discussione, sotto vari aspetti, i fondamenti del sentire comune dell'Unione europea, di questa che non è solamente una comunità politica, ma una comunità di popoli,

anche oggi da questo disegno di legge di delegazione europea può essere uno strumento, grande o piccolo che sia, di grandi o piccoli contenuti, che rappresenta però un tassello

l'annuale disegno di legge di delegazione europea, così come previsto dalla legge n. 234 del 2012, ha il compito principale di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo; un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Tale percorso passa attraverso fasi di negoziato gestite dal Governo, in cui la principale preoccupazione di chi se ne deve essere quella di tener conto dell'interesse nazionale delle nostre imprese, dei nostri cittadini e del nostro tessuto sociale ed economico. Le decisioni europee, infatti, in tutte le loro discutibili forme, incidono sulla vita politica, sociale ed economica del nostro Paese,

differente tassazione sul gioco d'azzardo; si parla dei veicoli degli studenti europei in Italia, delle aliquote IVA, del basilico, del rosmarino e della salvia freschi, dei tartufi e dell'indennizzo in favore delle vittime di reati internazionali violenti, di disposizioni relative alla natura della fauna selvatica; inoltre, il provvedimento reca raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e molto altro. argomenti sicuramente eterogenei, signora Presidente, di cui ricordiamo gli articoli 1, 2, 21, 22 e 23, che non sanano sanzioni ma ma intervengono sui casi EU Pilot che vanno a limitare i valori della trasparenza e correttezza delle informazioni. Questi articoli denotano infatti l'atteggiamento rinunciatario che questo Governo continua a tenere proprio nel settore agroalimentare, che dovrebbe invece costituire il vanto internazionale del nostro *made in Italy*.

volte ci siamo confrontati e a volte anche in modo piccato, ma sempre nella correttezza di chi cerca di portare del buono al proprio Paese. C'è però da dire che l'Europa come noi la intendiamo non è proprio questa. Noi vogliamo un'Europa che sia attenta ai cittadini, alle specificità dei propri territori, alla capacità di ogni Nazione di mettere in condizione i cittadini di trarre il meglio dalle capacità capacità che hanno sia sotto l'aspetto produttivo, che imprenditoriale. Una delle normative più balorde che abbiamo considerato in questo periodo è la direttiva Bolkestein, che non molti giorni fa non molti giorni fa ha determinato problematiche legate a chi sta gestendo i nostri litorali. Mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio che

forza e attenzione quando si è invitati a tre a un tavolo molto importante come quello successivo alla Brexit e al voto britannico: forse è il caso di capire che quell'invito è dovuto solamente al fatto che probabilmente, se un *referendum* di quel tipo fosse stato indetto in questo Paese, si sarebbe avuto lo stesso risultato. Il problema di questo Paese è molto semplice: non abbiamo un piano industriale, né energetico. Non abbiamo avuto neanche una strategia per il turismo...

finestra") *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi in Aula per discutere il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015». Noi tutti sappiamo che il disegno di legge di delegazione europea è composto complessivamente da deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei. Nessuno mette in dubbio l'importanza che ha questo disegno di legge, che darà attuazione nel territorio nazionale a numerose disposizioni dell'Unione europea e che avrà il compito di regolare diversi ambiti delle sfere economiche e sociali. Anche questa volta, però, come troppo spesso succede, ci troviamo a recepire norme dell'Unione europea in maniera compulsiva e automatizzata, senza avere il minimo scrupolo di approfondire le tematiche al loro interno e valutarne gli effetti che esse riverseranno in primo luogo sulla nostra legislazione e, di conseguenza, sulla vita di tutti i giorni dei cittadini italiani. L'appartenenza all'Unione europea non è in discussione, nessuno vuole mettere i bastoni tra le ruote agli obblighi che ci vengono impartiti per via della nostra adesione; quello che vogliamo è la possibilità di concordare questi obblighi. Chiediamo di avere la possibilità di redigere e negoziare, con le parti sociali e le categorie professionali chiamate in causa, quelle norme europee che avranno una loro influenza sui diritti intangibili e costituzionali garantiti. A tal proposito, mi sento di esprimere le mie paure e la mia perplessità su quello che ritengo essere il cammino intrapreso da questa Europa; un futuro in cui le tradizioni e le radici di ogni singolo popolo che la compongono sbiadiscono lentamente, fino a mischiarsi in una sorta di dio terreno e mortale, per citare il «Leviatano» di Hobbes, cui cediamo ogni nostro diritto naturale per garantirci, tramite la sua spada, la protezione da un non ben specificato nemico. Ma a differenza della società ipotizzata da Hobbes, le nostre culture, a partire da quella italiana, sono tutt'altro che composte da uomini solitari, poveri, pericolosi, brutali e dalla vita breve, e questo proprio grazie al dono prezioso dell'anima e della coscienza, da parte del Dio celeste ed immortale, al quale il Leviatano stesso deve sottostare. E siamo poi così sicuri che questo guerriero Leviatano sia effettivamente in grado di proteggerci? Se non abbiamo dei valori di riferimento, e nello specifico i valori più importanti ed innegabili, che sono proprio le nostre radici cristiane e la fratellanza in Cristo, quali istruzioni possiamo fornirgli per fargli discernere il bene dal male? Nessuna. Perché il concetto, semplificato, di bene e di male, sarà parametrato su un qualcosa di astratto, se non astruso, che con i valori non ha nulla a che vedere. «Una piccola cappella sulla via Appia Antica ci ricorda il nostro destino. Fu qui che, secondo la leggenda, San Pietro, mentre cercava di sfuggire alla persecuzione da parte delle autorità romane, fu fermato nella sua corsa dalla figura di Gesù, che gli apparve improvvisamente come spuntando fuori dal nulla. *Domine, quo vadis*? - domandò Pietro. Ma Gesù gli rispose facendogli la medesima domanda, e Pietro comprese che cosa doveva fare: tornò a Roma e portò a termine la sua missione». Questo scriveva, la bellezza di dieci anni fa, sir Roger Scruton, accademico e filosofo britannico, in un articolo intitolato proprio «*Quo vadis, Europa? Quo vadis, Italia?*». si interrogava sul fatto che, a parer suo, l'Europa stesse vivendo un tragico rifiuto di sé, aggiungendo che: «L'Europa sembra fuggire dal proprio passato, dalla propria eredità, dalla propria missione cristiana. Ma fugge senza avere una meta verso la quale dirigersi». Il grande progetto europeo, che dovrebbe giustificare tutti i mutamenti sociali, e politici che ci vengono imposti, ha improvvisamente perso la maschera e rivelato tutta la sua nullità. I politici hanno fatto calare questo progetto sulla nostra testa a forza di trucchi e di inganni. Gli Stati nazione dell'Europa, così ci hanno detto, resteranno liberi e democratici: vogliamo soltanto dare vita ad una riunione di amici, facilitare gli scambi commerciali e promuovere gli interessi comuni. Ma, poco a poco, la burocrazia è cresciuta, i nostri poteri legislativi ci sono stati sottratti e l'idea di lealtà nazionale è stata rifiutata e calpestata. Ma a quale scopo? Leggete la proposta di Costituzione europea e lo capirete. In nessun punto parla della religione dell'Europa, delle glorie e delle imprese del passato europeo o della grande cultura che il nostro Continente ha saputo produrre. Pagine e pagine di parole vuote, che rivelano una velata ostilità nei confronti dello Stato nazione; un'agenda politica sostanzialmente socialista, e una sistematica confisca dei poteri legislativi spettanti alle Nazioni. In questo documento non c'è nulla di chiaro, tranne quanto viene negato e rifiutato. Questo documento non è altro che un sistematico rinnegamento del passato europeo. I francesi e gli olandesi hanno votato contro questa proposta di Costituzione (e, aggiungo io, nel lontano 2005). Ma questo non significa che verrà abbandonata. Il progetto europeo è uguale al progetto bolscevico del 1917: non c'è alcun piano B. La macchina è stata messa in moto; e quando è deragliata, gli ingegneri l'hanno semplicemente rimessa sui binari. Ogni tanto i politici parlano di un "percorso lento" e di un "percorso veloce'' per il futuro; ma portano entrambi nella stessa direzione: vale a dire, da nessuna parte. Alla data attuale, tanto per capire quanto queste speculazioni hanno colto nel segno, il Regno Unito è uscito dall'Unione europea, portandosi appresso il malumore di tanti altri Paesi, evidentemente costretti senza troppa convinzione ad abbracciare questo progetto. Tornando ad esaminare il provvedimento in questione, esso è stato approvato alla Camera dei deputati in prima lettura con 314 voti favorevoli e 80 contrari ed è stato presentato dal Governo il 18 gennaio 2016. Molteplici modifiche e integrazioni sono state apportate, durante l'esame parlamentare, al testo iniziale del disegno di legge di delegazione europea 2015. Le novità vertono principalmente sull'introduzione di principi e criteri specifici di delega per il recepimento di diversi atti dell'Unione europea e l'introduzione di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea da rendere operativi nell'ordinamento nazionale. Il provvedimento approvato alla Camera si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto 12 direttive europee, CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), una decisione quadro, e infine l'adeguamento delle normative nazionale a 13 regolamenti europei. Il Governo è stato autorizzato al recepimento delle direttive sull'equipaggiamento marittimo e della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana in via regolamentare. Sono state apportate considerevoli integrazioni al contenuto del disegno di legge governativo originario, utilizzando principi e criteri di delega e l'inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

dal fare una valutazione di caratura politica su quella che è oggi l'Unione europea e quello che è diventato questo rituale di modifica del nostro modo di vivere e della nostra legislazione in funzione delle direttive europee. da troppo tempo che ci stiamo abituando a recepire qualsiasi cosa venga dall'Unione europea in termini

sul significato dell'appartenenza all'Unione europea. Infatti, se un significato bisogna o si può trovare, credo che questo non possa essere nel mero recepimento di direttive o regolamenti che riguardano la riduzione dell'utilizzo delle borse in plastica o in materiale leggero, piuttosto che misure di coordinamento per la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea o, ancora, altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame, come la definizione dei termini

Tutto ciò appare invece totalmente estraneo al dibattito. Perché? Certamente da parte dell'Italia c'è ormai da troppo tempo una posizione di passività nei confronti dell'Unione europea, che porta a rinunciare alla difesa degli interessi propri dei nostri cittadini e delle attività produttive.

alla Commissione europea una risoluzione che terminava con l'auspicio della centralità dei negoziati di adesione con la Turchia, cui l'Italia è fortemente favorevole:

tale risoluzione si scriveva: «La 14a Commissione ribadisce infine l'importanza della Turchia sul piano economico e strategico, soprattutto nel suo ruolo di elemento di stabilità e per l'equilibrio geopolitico dei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente». Che lunga visione! «Nel ribadire il sostegno alla prospettiva europea, sottolinea tuttavia non senza preoccupazione l'impatto che gli eventi di maggio e giugno 2013 a Istanbul rischiano di esercitare sul processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche e di apertura alle istanze della società civile, e auspica che il e auspica che il Governo turco stigmatizzi con forza l'uso della violenza contro qualunque manifestazione di protesta

Stiamo cadendo nel ridicolo, perché si sta parlando di provvedimenti dell'Unione europea e si trascura totalmente lo scenario nel quale l'Unione europea in questo momento si sta dissolvendo. Noi oggi siamo chiamati dal relatore

il Regno Unito è uscito dall'Unione europea qualche settimana fa e che il nostro Paese si è espresso con applausi e ampio sostegno nei confronti dell'ingresso della Turchia in Europa. stessa Turchia che, in questi giorni e in queste ore, sta riempiendo non le galere, ma i campi di concentramento di cittadini rei di avere una posizione politica di dissenso rispetto al dittatore Erdogan, cui la stessa Unione europea ha appena elargito 3 miliardi di euro per fargli gestire i confini d'Europa. Non occorre avere grande fantasia per ricordare che il grande momento di decadenza dell'Impero romano avvenne nel momento in cui i romani pagarono le truppe per mantenere la pace ai confini. Questo è quello che sta accadendo oggi. L'Unione europea, da una parte, viene vissuta come recepimento di normative sui sacchetti per la spesa dall'altra, paga i mercenari al confine e chiude gli occhi rispetto a Governi, come quello turco, che prendono la prima opportunità - la storia ci racconterà cosa stava dietro questo *golpe* fallito - per fare repressione contro la democrazia nel Paese. In silenzio e in connivenza l'Unione europea manda qualche dispaccio e piccola rimostranza, ma ben si guarda dal prendere netta posizione contro questa situazione. Questo darebbe un significato alla nostra partecipazione all'Unione europea e non il recepire normative che riguardano le buste per andare a fare la spesa al supermercato. Se oggi dobbiamo parlare di cose serie, dobbiamo ricordarci che la nostra partecipazione all'Unione europea ha comportato il *bail in* significa aver messo sul lastrico decine di migliaia di famiglie per aver recepito una normativa in maniera acritica acritica per parte di maggioranza. Noi, quando fu il momento, dicemmo di fare attenzione perché queste stesse regole, applicate in Italia e con un sistema come il nostro, avrebbero avuto effetti devastanti rispetto a quanto ha fatto la Germania anzitempo sistemando i conti delle proprie banche

Vedremo adesso, in fase di esame degli emendamenti, quale sarà l'atteggiamento del Governo. Ci compiacciamo del fatto che in Commissione siano stati recepiti molti nostri ordini del giorno; ma ci dispiace che la Commissione non abbia recepito alcun emendamento, per la volontà di non modificare il provvedimento al Senato. a concludere - hanno bisogno che il Governo, prima di attuare e di recepire le direttive europee, consideri la loro ricaduta nei confronti di chi il mondo lo vive nella realtà, perché troppo spesso si recepiscono le direttive europee solo per non andare in infrazione, trascurando il fatto che poi queste normative devono essere applicate. E i cittadini, spesso e volentieri, si trovano ad avere a che fare con una burocrazia già troppo soccombente. Su queste cose vogliamo che si faccia la differenza; aspettiamo la fase emendativa per esprimere un giudizio.

di un provvedimento delicato ed importante, in virtù della sua natura di strumento di adeguamento di quanto produciamo in Italia dal punto di vista legislativo di ciò che vorrebbe - vuole - l'Unione europea, in tutte le materie, dall'agricoltura all'industria, ai servizi del terziario, al commercio. È un processo che appare particolarmente difficoltoso e traumatico per il nostro Paese, in quanto la scarsa incisività dell'Italia a livello istituzionale nelle sedi giuste e nei momenti giusti, determina una scarsa capacità di tutelare e salvaguardare gli interessi del Paese in quelle sedi e fa sì che ogni anno il Parlamento e il Governo si trovino ad emanare leggi ed atti con forza di legge, spesso molto in ritardo rispetto alle scadenze europee, sotto la minaccia dell'avvio di nuove procedure di infrazione. Come tutti sappiamo, questo fa sì che il nostro ordinamento si trovi ad essere letteralmente invaso da norme di difficile inserimento, quando non completamente contrastanti con principi ed interessi importanti per la nostra società. Il presente disegno di legge fa emergere chiaramente che non siamo stati sufficientemente presenti nella fase ascendente della produzione legislativa europea. Inoltre, il Governo è stato anche poco attento ad adottare misure e comportamenti che avrebbero potuto mitigare l'impatto

la consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, comportamento che invece dovrebbe essere di primario interesse al fine di studiare, di concerto con tali associazioni portatrici di legittimi interessi, le soluzioni più idonee a tutelare gli interessi dei cittadini e della Nazione. Per esempio, proprio su questo punto all'articolo 20 del provvedimento, il quale stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva europea n. 26 del 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore

interpellare le associazioni di settore, che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa. Inoltre, è stata è stata sottolineata la necessità che, prima dell'esercizio della delega, il Governo provveda a definire in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva (sempre sui diritti d'autore), in ossequio all'articolo 8 della direttiva la quale stabilisce una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri. Riguardo all'articolo 5, con cui si delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché di adeguarla a quella sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, ho presentato alcuni emendamenti, vista la rilevanza di questa tematica per il nostro settore agroalimentare, troppo spesso vessato e mortificato dalle politiche comunitarie che, tardi, troppo tardi, hanno scoperto che in Italia e negli altri Stati nazionali la biodiversità e i processi tradizionali produttivi e le tipicità sono valori e vanno tutelati. tutelati. L'emendamento 5.7 persegue il fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui anche oli extravergini di oliva, a denominazione di origine protetta (DOP),

per i quali abbiamo proposto che le modalità per l'integrazione dell'etichettatura fosse realizzata con sistemi di sicurezza predisposti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, basati su elementi elettronici o telematici. ciò per ridurre considerevolmente il rischio di contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio, L'articolo 12 del provvedimento stabilisce i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione della direttiva n.

poiché i proventi di tali sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato, l'emendamento 12.4 propone di destinarli al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Infine, a nome a nome dei Conservatori e Riformisti, abbiamo proposto anche un intervento più chirurgico nell'emendamento 12.5, che prevede la possibilità di valutare che i proventi confluiscano, per il 50 per cento, al Fondo interbancario di tutela dei depositi, che a sua volta alimenta il Fondo di solidarietà istituito dal comma 856 della legge di stabilità e destinato al risarcimento degli obbligazionisti delle quattro banche liquidate per il triennio 2017-2019 e per il 50 per cento alla riduzione della pressione fiscale, mentre dal 2020 al solo fondo per la riduzione della pressione fiscale. è chiaro che occorre utilizzare questa occasione di dibattito in Parlamento, fra Commissione ed Assemblea, per determinare un *focus* sul funzionamento delle regole e sullo spirito comunitario dell'Unione. Tutto ciò che sta accadendo in Europa, a cominciare dalla Brexit, deve aprirci occhi ed orecchi sulle ragioni dell'Unione e verificare la validità dello stare insieme e la percezione popolare delle funzioni nelle Grazie,

inadatti a risollevare lo Stato da questa crisi prociclica, emblema di una Europa che sa solo sanzionare senza tener conto degli effetti sui cittadini. che addirittura ora impone persino di autosanzionarci, di trovare le sanzioni a noi più consone in caso di violazioni degli obblighi contenuti nelle direttive europee, dando carta bianca per nuove fattispecie di reati e illeciti amministrativi. Sto parlando dell'articolo 2 e del fondo di 100 milioni l'anno per le sanzioni. In pratica, ci autosanzioniamo e distogliamo patrimonio che potrebbe essere destinato al sociale. Dalla lettura della suddetta legge sembra che l'Italia si appresti a recepire tutta una serie di provvedimenti che da qui a poco ci faranno pensare che il peggio sia passato. Eppure io non vedo altro che cornici vuote e profonde contraddizioni. In particolare mi sono soffermata sulle sanzioni e sugli accorgimenti per evitare il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per praticare la tortura, infliggere la pena di morte e altri trattamenti o pene crudeli e degradanti. Mi sembra, però, un provvedimento che non vada a contrastare il fatto dell'assistere ad una sempre maggiore corsa agli armamenti nucleari: congegni ogni giorno più sofisticati e distruttivi. Non si tratta forse di strumenti capaci di procurare la morte? L'Italia è divenuta un gigantesco arsenale per missioni militari offensive ed invasive in nome di una neutralità soltanto dichiarata e mai praticata. Senza contare che il nostro Stato esporta e vende armi verso Paesi che violano diritti umani o comunque verso aree di conflitto. Si tratta nella maggior parte di "Paesi amici" con cui intratteniamo rapporti commerciali. Come rifiutarsi quindi? Anche se questo significa porre in pericolo intere popolazioni potenzialmente soggette a pena di morte, tortura e pene degradanti,

esportazioni destinate anche a Paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Iraq, Arabia Saudita, Pakistan, sono solo alcuni dei Paesi verso i quali c'è stata l'impennata di esportazioni di armamenti come razzi, agenti tossici e chimici e via discorrendo. In particolare le esportazioni verso la Turchia sono passate da 53 a 129 milioni di euro. D'altronde non scordiamoci che questa Unione europea si è resa protagonista di ingenti stanziamenti di risorse verso la Turchia, luogo in cui le guardie di confine sparano sui profughi, lasciando Ankara bombardare indisturbata il popolo curdo. Per quanto riguarda, poi, il tema degli embarghi commerciali, vorrei sottolineare che le sanzioni contro la Russia introdotte dall'Unione europea sono costate all'Italia 3,6 miliardi di euro di *export* che riguarda soprattutto il settore manifatturiero in un periodo di profonda crisi industriale italiana che assiste ogni giorno ad un gran numero di delocalizzazioni ad opera delle multinazionali con ingenti perdite dei posti di lavoro. Insomma davvero una brutta batosta per il *made in Italy*. In generale non posso condividere le posizioni di una Unione europea così strutturata, basata sul continuo aumento dell'influenza e del potere che i grandi monopoli hanno nell'economia e nel condizionamento politico degli Stati. Di una Unione europea che, nella realtà dei fatti, benché si appresti a tutelare i consumatori riguardo alle diciture o marche che consentono di identificare la partita la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, rappresenta la pietra tombale del settore agricolo italiano a beneficio della circolazione di merci a bassissimi costi e di qualità scadente e a discapito delle coltivazioni tradizionali e radicate che hanno cessato di essere produttive. Unione europea cerca di arginare, sulla carta, l'inquinamento atmosferico e poi nei fatti non presta attenzione alla letteratura internazionale sulle fonti rinnovabili, facendo ricadere in questa accezione anche fonti di energia estremamente inquinanti, suggellandole con ingenti con ingenti incentivi. Un'Europa che si dice attenta agli interessi e alla protezione dei consumatori e risparmiatori e poi detta dall'alto come risoluzione bancaria il *bail in* che ha creato il panico fra i risparmiatori senza contarne l'incostituzionalità per contrasto con l'articolo 47 della nostra Costituzione che tutela il risparmio sotto ogni forma. Per queste e molte altre considerazioni che ci sarebbero da mi sento di assumere ancora una volta una posizione di critica e contrasto verso i provvedimenti europei da recepire. *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sulla parte di questo disegno di legge, l'articolo 20, che si riferisce alla tutela e all'esercizio dei diritti d'autore.

la libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore da parte dei titolari dei diritti stessi. A questo proposito l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nel parere del 1° giugno scorso, ha avvertito il Parlamento e il Governo, in modo molto netto, molto netto, che «il valore e la *ratio* stessa dell'impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza,

che attribuisce a un solo soggetto (SIAE) la riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore». Dunque, un rilievo molto *tranchant*,

del mercato nazionale della gestione dei diritti d'autore limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'*incumbent* senza discriminazioni». La necessità che questo disegno di legge, ormai in seconda lettura, venisse approvato immediatamente senza emendamenti

sul presupposto dell'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità dalla Commissione e che è stato richiamato dal relatore in apertura di questa discussione. L'ordine del giorno impegna il Governo, in modo molto preciso, «a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti» - dalla norma così com'è, che però l'Antitrust ci avverte essere insufficientemente attuativa del contenuto della direttiva - «in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione

un impegno molto preciso che deve portare in tempi brevi al superamento dell'attuale regime di monopolio. Questo è l'unico modo in cui possiamo superare le gravissime inefficienze - ma io direi anche anomalie

può mantenere oggi una struttura gravemente ipertrofica, costosissima: costa il doppio del CNEL; è un costo che viene ribaltato con gli stessi

stampa ed emittenti televisive di vario segno, circa la gestione delle migliaia di dipendenti di questa struttura, appunto, in termini di clientelismo e nepotismo. Si tratta, soprattutto, di una struttura incapace di garantire la trasparenza richiesta dalla direttiva, sia nel processo di esazione del diritto d'autore da chi utilizza l'opera artistica, sia soprattutto nella distribuzione del provento a chi ne ha dritto. Oggi i criteri di distribuzione ai titolari del diritto d'autore sono assolutamente

Concludo con l'auspicio che l'impegno assunto dal Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno, che viene riproposto in Assemblea come ordine del giorno della Commissione G20.101

questa sede - ad accogliere e attuare le indicazioni contenute nel parere dell'Autorità *antitrust*, venga onorato in modo compiuto e puntuale, così voltandosi pagina rispetto a una lunga stagione segnata dal regime di monopolio, che sta penalizzando in modo grave l'attività letteraria e artistica nel nostro Paese.

Presidente, colleghe e colleghi, partendo dalla considerazione che il Senato ha esaminato la legge europea e la Camera ha esitato senza variazioni il nostro testo, altrettanto pare avverrà per il disegno di legge di delegazione europea arrivato dalla Camera, che il Senato si appresta a votare tal quale. Grazie,

per ciò che sta avvenendo in Italia, dove intere categorie manifestano perplessità sull'appartenenza alla Comunità europea. È di oggi la notizia di una forte protesta nel mondo agricolo - parlo dei produttori di grano che sostengono che il grano non dà pane. Crolla il prezzo del grano, Coldiretti Confagricoltura (stranamente insieme), CIA e Coopagri scendono in piazza per protestare, lamentando che il prezzo è sceso quasi al minimo storico, ovvero a quello di cinquant'anni fa,

ovvero indicazioni sulla qualità del prodotto, ovvero ancora la dicitura *made in Italy*. È su questo riconoscimento che la considerazione diventa di carattere politico. La UE infatti nega questo riconoscimento, che più volte è stato richiesto, ma non siamo mai riusciti ad ottenere un'apertura, non siamo mai riusciti ad ottenere un marchio che assicuri il consumatore, favorendo la produzione italiana che in molti settori è di qualità indubbiamente superiore. Oggi stiamo parlando del grano, ieri abbiamo parlato dell'olio,

di tante altre cose. Mi chiedo come si faccia a convincere queste categorie, che rappresentano un asse portante anche della nostra economia, a dire che l'appartenenza all'Europa crea loro vantaggi. Certo, il *made in Italy* risente della debolezza politica dell'Italia in seno alla Unione europea origina la mia seconda riflessione. L'Italia, quale Stato fondatore, non gode del ruolo che dovrebbe esserle riconosciuto

che ha convocato la Germania, la Francia e l'Irlanda per discutere su temi importanti, tra cui quelli ufficiali come i tempi di uscita e di scrittura dei trattati di cooperazione del dopo Brexit.

tra i quali considero anche importante il rafforzamento dello spirito di appartenenza all'Unione europea. È vero che siamo in attesa del *referendum*,

competenza sarà destinato il nuovo Senato, laddove i senatori nuovi eletti o nominati abbiano da svolgere un doppio ruolo: quello di sindaco o consigliere regionale e, contemporaneamente, quello di senatore. Mi spaventa veramente pensare che queste persone, seppure di intelligenza superiore, abbiano più tempo da dedicare alla 14a Commissione

Grazie,

in relazione all'articolo 2635 del codice civile in materia di corruzione tra privati, fattispecie riservata alle infedeltà rispetto agli obblighi d'ufficio, dei vertici aziendali, sindaci o revisori, qualora cagionino nocumento all'azienda, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità. L'articolo 19 introdotto dalla Camera intende dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella decisione quadro del 2003, n. 568, GAI per la disciplina del reato di corruzione tra privati, tassello di un *puzzle* di contrasto a un fenomeno più ampio e generalmente collegato ai reati contro la pubblica amministrazione; fenomeno che mina le regole della concorrenza nel mercato interno e dell'economia legale, contrasto alla corruzione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e a tutela dei diritti dei singoli imprenditori; fenomeno corruttivo che indubbiamente lede un bene più generale, che è quello della integrità del funzionamento dello Stato di diritto, mina la democrazia e le regole del vivere comunitario. È un fenomeno, la corruzione, che, oltre a sottrarre risorse al ciclo dell'economia reale e alle opportunità di occupazione, scoraggia e allontana investimenti esterni e quindi potenzialità di crescita, perché rompe il rapporto di fiducia che lega cittadini, imprese e Stato, alimenta la percezione di diffusa diffidenza, mina la coesione sociale ed economica. Tale rilievo ha portato con la decisione quadro del 2002, n. 584, relativa al mandato di arresto europeo, a includere la corruzione nell'elenco dei reati in relazione ai quali non è richiesta la verifica preliminare della doppia incriminazione ai fini dell'applicazione della misura. Particolarmente importante, in tale quadro, è pertanto arrivare alla determinazione di norme minime comuni di definizione della stessa fattispecie penale, perseguibile in tutti i Paesi membri, oggi ancora mancante. Il Consiglio d'Europa, con l'approvazione della Convenzione penale sulla corruzione nel 1999, ha istituito con uno specifico protocollo un gruppo di Stati, il gruppo "Greco", per l'individuazione delle buone pratiche di lotta a tale fenomeno corruttivo, sia pubblico che privato. Proprio nella terza relazione del gruppo "Greco" nel 2012 veniva evidenziato come il fenomeno della corruzione tra privati sia percepito come meno diffuso e meno grave e come in Italia non ci fosse a quella data nessuna effettiva applicazione delle disposizioni dell'articolo delle disposizioni dell'articolo 2635 del codice civile, introdotto nel 2002, non registrando alcuna incriminazione ai sensi di tale norma. Garantire, pertanto, una effettiva ed efficace perseguibilità delle condotte di corruzione privata, come statuito nella decisione del 2003 di cui la legge di delegazione completa l'attuazione, rappresenta una priorità, per includere nella fattispecie incriminatoria sia condotte attive che passive, estendendo la responsabilità alle persone giuridiche che beneficiano di tali atti corruttivi, persone giuridiche a fine di lucro, ma anche persone giuridiche senza scopo di lucro. lucro. Il mirino di tale lotta va, infatti, puntato sulla cultura stessa della corruzione, che può manifestarsi tanto nel settore economico privato, quanto nella pubblica amministrazione. Più in particolare, la decisione quadro invita gli Stati ad adottare misure per assicurare che condotte intenzionali costituiscano illecito penale se compiute nell'ambito di attività professionali, condotte di istigazione e favoreggiamento, istigazione privata che superi la previsione di cui all'articolo 414 del codice penale, prevedendo anche la procedibilità d'ufficio, nonché sanzioni proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche responsabili, comprese pene accessorie interdittive quali il divieto di esercizio temporaneo di attività. Una specifica e significativa pena accessoria potrebbe essere inserita, e nel nostro ordinamento potrebbe fungere da deterrente effettivo e costituirebbe misura di giustizia, ovvero l'esclusione dell'azienda responsabile di corruzione dagli aiuti pubblici, dagli aiuti di Stato e ogni altra forma di sostegno economico o finanziario pubblico. La completa attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 19 consentirebbe, infine, di risolvere una procedura della Commissione europea EU *pilot* del 2015 per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro del 2003, per completare la previsione della legge Severino (legge n. 190 del 2012) della punibilità per corruzione privata anche per chi avanzi la richiesta di un vantaggio indebito; corruzione tra privati, in violazione dei propri doveri a tutela di un bene che è espressione della lealtà e fiducia, indispensabile per sane relazioni professionali tra privati come nel settore pubblico, sintomo e misura del grado di senso civico, del rispetto delle regole scritte ma anche morali ed etiche che la convivenza civile impone perché il danno è prodotto anche quando non si rilevi una perdita effettiva per l'azienda, ma solo per aver generato un rapporto corruttivo in violazione delle regole di concorrenza leale. Lotta all'economia deviata e illegale contro cui in questi due anni abbiamo definito nuovi strumenti di contrasto, dal rafforzamento dei poteri dell'ANAC, all'introduzione del reato di autoriciclaggio, all'inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione e con la reintroduzione della fattispecie penale di reato delle false dichiarazioni L'Unione europea con il Trattato di Lisbona si è posta l'obiettivo ambizioso di arrivare a creare uno spazio di libertà sicurezza e giustizia unico; un obiettivo che comporta determinazione nel definire nuovi ed efficaci strumenti di contrasto a gravi fenomeni, quali il terrorismo, la gestione dell'immigrazione e l'asilo, la lotta alla criminalità e alle frodi, compresa la corruzione, così come indicato nel pacchetto anticorruzione presentato dalla Commissione europea nel 2011. tasselli che costituiscono di fatto i mattoni su cui poggiare le fondamenta di quella nuova Europa unita che tutti invocano e che da ieri siamo stati chiamati a costruire in maniera più celere, più stretta, ma anche più rigorosa in termini di legalità; più democratica, più vicina ai cittadini e più attenta a consegnare alle future generazioni una unione più giusta ma soprattutto più sicura.

Signora Presidente, pochi giorni fa ho incontrato una delegazione di lavoratori delle ex Acciaierie Lucchini di Piombino e dell'indotto che si sono raccolti e associati nel Coordinamento articolo 1 - Camping CIG. Questi lavoratori si sono uniti in un Coordinamento per tutelare il proprio diritto al lavoro, messo sempre più in discussione da politiche del lavoro e industriali sbagliate e dall'assenza di un intervento deciso e chiaro da parte delle istituzioni e dei sindacati. Le acciaierie di Piombino negli ultimi anni sono passate dalla gestione della famiglia Lucchini alla società russa Severstal, fino ad arrivare all'acquisizione degli algerini di Cevital. In data 11 marzo 2015 avevo già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03838, presso il Ministero dello sviluppo economico, in cui avevo chiesto accesso completo agli atti riguardanti l'accordo tra Governo e Cevital. Tuttavia, questa richiesta non ha mai avuto risposta. Ormai abbiamo capito che avere risposte da questo Governo è quasi impossibile, come vincere alla lotteria! Ricordo che l'accordo, firmato tra il presidente della società Cevital, Issad Rebrab, e il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino, signor Piero Nardi, a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente Renzi, del Ministro dello sviluppo economico, del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e del sindaco di Piombino ebbe una grande, grandissima rilevanza mediatica. Il presidente Renzi dichiarò: «Esprimo gioia, soddisfazione e gratitudine perché questo è l'accordo strategico che rappresenta un grande messaggio agli investitori stranieri

basano tutti gli accordi finora sottoscritti, non è mai stato realizzato. In secondo luogo, la procedura di verifica della necessità del VIA si basa su un piano industriale ridotto e, dunque, vi è la prospettiva certa che non tutti i lavoratori è alcuna sicurezza sui finanziamenti né per il circolante, né per gli investimenti. Anche se Cevital realizzasse il piano industriale, seppur in versione ridotta, lo stabilimento di Piombino non avrebbe un futuro certo senza il varo di un piano nazionale della siderurgia, che permetta di mettere in sinergia i vari siti siderurgici e che promuova la ricerca per giungere a prodotti di qualità sempre più alta. Infine, rimangono forti dubbi su quello che accadrà il 1° luglio 2107, quando Aferpi non avrà più gli obblighi di legge a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali

Grazie,